recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, premesso che:

Il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 6, interviene sull'organico della Corte di cassazione per potenziarlo e consentire il mantenimento in servizio dei vertici; modifica il procedimento in Cassazione; introduce misure di efficienza per gli uffici giudiziari, volte principalmente a garantire la celere copertura degli uffici vacanti; introduce misure per potenziare gli uffici di sorveglianza. Più nel dettaglio, l'articolo 1, introducendo due ulteriori commi all'articolo 115 del regio decreto n. 12 del 1941, prevede che i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, che sono magistrati con funzioni di merito, possano essere impiegati eccezionalmente per comporre i collegi giudicanti, tanto civili quanto penali, della Corte di cassazione al fine di rafforzare i presidi organizzativi necessari a un più rapido smaltimento dell'arretrato. L'applicazione temporanea dovrà essere disposta tenuto conto delle tabelle di organizzazione della Corte e delle esigenze dell'Ufficio del massimario. L'articolo nella sua formulazione originaria circoscriveva la possibilità di svolgere funzioni giurisdizionali di legittimità ai magistrati che avessero presso l'Ufficio del massimario un'anzianità di servizio di almeno due anni;

e ponendo un limite triennale (non rinnovabile) all'applicazione. Il nuovo articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, la Camera, reca numerose modifiche al procedimento di Cassazione. Tali modifiche ricalcano sostanzialmente il contenuto dei principi di delega previsti dall'articolo 1, 2, lettera c) dell'Atto Senato 2284, (Delega per la riforma del processo civile), già approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione giustizia. In particolare, il comma 1 della disposizione generalizza l'uso della trattazione in camera di consiglio nei procedimenti civili che si svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte e modifica la procedura del cosiddetto filtro in Cassazione. Il comma 2 dell'articolo 1-*bis* reca una disposizione transitoria prevedendo che la riforma del procedimento di cassazione si applichi ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e ai ricorsi per i quali non è stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio. L'articolo 2, al comma 1, modificando l'articolo 73 del decreto-legge 69 del 2013, estende la previsione di tirocini formativi presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la Corte di cassazione, stabilendo che l'attività di formazione degli ammessi allo *stage* sia condotta in collaborazione con il Consiglio nazionale forense, nonché con le scuole di specializzazione per le professioni legali. I commi da 2 a 5 dell'articolo 2 intervengono sulla disciplina del concorso per magistrato ordinario, consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero di posti banditi a concorso, in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici, e riducendo in via eccezionale, da diciotto a dodici mesi, la durata del tirocinio dei magistrati che saranno nominati a seguito dei concorsi già banditi (nel 2014 e nel 2015), per consentire loro di svolgere quanto prima le funzioni giudiziarie; è fatta eccezione per i magistrati vincitori del concorso riservato alla Provincia autonoma di Bolzano, nominati a fine 2015. La Camera è intervenuta sul comma 3 per ridurre a un mese la durata del tirocinio teorico presso la Scuola superiore della magistratura (il decreto-legge prevedeva due mesi) e conseguentemente ampliare a undici mesi (in luogo dei previsti dieci) il tirocinio presso gli uffici giudiziari. L'articolo 3 reca disposizioni

termine di tre anni) nella sede precedente. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato precisato che queste disposizioni non si applicano Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato precisato che queste disposizioni non si applicano né ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto legge,

al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale della medesima Corte, prevede il trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2017, per coloro che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra lo predetta data e il 30 dicembre 2017 L'articolo 6 interviene sul ruolo organico della magistratura ordinaria per ridurre di 52 unità i magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado e aumentare in misura corrispondente il numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e secondo grado L'articolo 7 modifica alcune disposizioni del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 relative al domicilio digitale, alla possibile deroga alla regola del deposito telematico degli atti processuali e alla copie informatiche degli atti processuali.

il ricorso e gli altri atti processuali nel rispetto di limiti dimensionali che saranno dettati da decreti del Presidente del Consiglio di Stato, all'esito di un procedura di consultazione delle categorie di professionisti interessate, entro la fine di quest'anno. L'articolo 8 del decreto-legge istituisce l'ufficio per il processo amministrativo sulla falsariga del modello introdotto nella giustizia ordinaria. L'articolo 9 reca disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa, prevedendo un aumento totale di 53 unità di personale, da assumere con contratto a tempo indeterminato mediante concorso pubblico L'articolo 10 disciplina la proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato negli stessi termini enunciati per i magistrati ordinari. Infine, il Capo III, composto dagli articoli 11 e 12, reca le disposizioni finanziarie e finali. Nella seduta del 12 ottobre la 1a Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo, con rilievi riferiti agli articoli 5 e 10, che si riporta in allegato. Il dibattito in Commissione giustizia - si è svolto nelle sedute pomeridiana e notturna dell'11 ottobre, nella seduta del 12 ottobre e in quelle pomeridiana e notturna del 17 ottobre - si è incentrato prevalentemente sugli articoli 1, 1-*bis*, 3,

i rilievi per i quali sarebbe opportuno non procedere all'esame del disegno di legge di conversione

che attengono alla violazione sia del principio del diritto di difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione, nonché di altre norme della Carta dei diritti per quanto riguarda la regolamentazioni dei ruoli e delle funzioni della magistratura. Mi riferisco agli articoli 5 e 10 del disegno di legge che, sulla scia di una proroga alla terza in materia di età per il pensionamento dei magistrati italiani - dispongono solamente per alcune cariche apicali della magistratura ordinaria, contabile e amministrativa

riguarda solamente le cariche apicali della Corte di cassazione e, mantenendo il limite di età a settanta anni, anche i vertici della giustizia amministrativa e contabile.

comporta un'evidente disparità di trattamento nell'ambito dei ruoli della magistratura, poiché espropria il Consiglio superiore della magistratura del suo compito, costituzionalmente previsto, di disporre le assunzioni e le assegnazioni.

pur essendo formalmente non ostativo - ci rendiamo conto degli equilibrismi a cui la maggioranza deve ricorrere, ma è da leggere - e rilevando le medesime criticità cui facevo riferimento,

che dovrebbero far gridare allo scandalo e alla necessità di abbandonare un ruolo politico che evidentemente questo Governo non sarebbe in grado di mantenere, dovendo ricorrere in maniera così sistematica alla forzatura del voto di fiducia, tanto più se in materia di giustizia e di magistrati, di giustizia e di magistrati, e che ci consegnerebbe uno dei periodi più bui della storia parlamentare. Vi sono poi altri profili di illegittimità costituzionale, come l'introduzione, nell'articolo 1-*bis*, di una violazione

ad affrontare al buio una possibile dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Mentre adesso una statuizione di inammissibilità o di manifesta infondatezza di un ricorso per Cassazione può essere oggetto di verifica nell'ambito degli uffici della Suprema corte, nel testo vigente scompare l'inciso ove si prevede che il presidente della sezione, seppure in maniera concisa, esponga le motivazioni in virtù delle quali, in camera di consiglio, si discuterà di una possibile dichiarazione di inammissibilità. Ebbene, questo inciso scompare e rimangono come dei simulacri le possibilità da parte dei difensori di rassegnare memorie entro cinque giorni prima dell'udienza. Ma capite bene che rassegnare memorie su cui esporre una tesi contraria sarà un richiamo assolutamente vuoto, perché non si conosceranno le motivazioni in virtù delle quali vi è stata una prima valutazione di inammissibilità. Questo chiaramente significa scoraggiare e non voler risolvere i problemi i problemi del carico giudiziario, in questo caso della Corte di cassazione, ancora una volta - e secondo una tradizione che ormai si perpetua da anni - scalciando via il cittadino e la tutela dei suoi diritti.

un numero di pagine che sarà determinato successivamente. Neanche Rabelais, che nel Cinquecento ha stigmatizzato satiricamente certa giustizia sommaria, con la figura del giudice che decideva tirando i dadi, tanto più piccoli quanto più complicata fosse la materia, avrebbe mai anche solo immaginato una simile aberrazione. Approvare una tale norma è la morte di ogni processo giusto; è la negazione della possibilità di far valere, davanti a un giudice imparziale, i propri interessi legittimi e i diritti soggettivi.

ugualmente non urgente riforma del procedimento davanti alla Cassazione civile, cui ho fatto riferimento prima. Quindi, le motivazioni che impongono la dichiarazione di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2550 ci appaiono ci appaiono solide. Non vi rendete complici. Siccome io dico no a titolo personale, da cittadino e da membro di questo Gruppo politico, ormai i nostri inviti cadono nel vuoto ed è inutile invitare, dico semplicemente no. Non fate un ulteriore scempio alla giustizia e diciamo no tutti insieme.

abbiamo presentato la questione pregiudiziale di costituzionalità al nostro esame nella speranza che vi sia un rinsavimento del Governo e della maggioranza.

di miglioramento del testo in senso costituzionale, in modo da evitare che norme necessarie possano poi essere caducate dalla Corte costituzionale. Un qualsiasi giudice, infatti, nell'applicare le leggi sceglie la norma e l'interpretazione più coerenti con la Costituzione. Un legislatore, quindi, quando ha la possibilità di correggere e rendere costituzionalmente corretta una norma, ha l'obbligo di provvedere. Mi limiterò soltanto ad alcuni aspetti:

non vi è dubbio che è incoerente con l'argomento del decreto. Eppure, ci siamo limitati a presentare due emendamenti - mi rivolgo proprio a lei, signor sottosegretario Migliore

l'articolo 3, esso contiene un errore che rende incostituzionale la norma. Vi siete resi conto alla Camera che vi era la necessità di garantire, con una norma transitoria, che chi aveva già maturato i tre anni come uditore giudiziario fosse legittimato rispetto al previsto aumento del periodo di legittimazione, Vi rendete conto che questo determina un'incoerenza e un contrasto forte con magistrati che hanno anni in più e hanno già maturato i tre anni? In questo caso creereste un privilegio e uno squilibrio all'interno della magistratura, a causa della disparità di trattamento.

non risponde e non spiega perché non accoglie un emendamento del genere. una norma che altera, all'interno del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l'equilibrio tra i magistrati del TAR e i magistrati del Consiglio di Stato. Stato. Abbiamo presentato un emendamento che rende coerente la norma con i principi della Costituzione con quell'equilibrio, ma non abbiamo avuto risposta.

dell'intelligenza politica della presidente Finocchiaro che ha portato a due affermazioni coerenti. In primo luogo, l'attuale testo certamente presenta profili di incostituzionalità

chiusura della età pensionabile dei magistrati, una diversa realtà. Calare una norma del genere nella pubblica amministrazione è possibile. Non è possibile nella magistratura, nei confronti di chi amministra la giurisdizione. O siete incompetenti o non vi rendete conto. L'anno scorso avete fatto una proroga che era corretta: non creava disparità di trattamento e riguardava solo gli uffici direttivi e i semi direttivi. Signori Sottosegretario e relatore, abbiamo presentato due emendamenti: uno ripete la stessa proroga dell'anno scorso, risolvendo anche, rispetto alla proroga degli uffici direttivi (sono non molti, come sapete, ma pochissimi,

coerente con il principio di dover svolgere la nostra funzione nell'interesse generale del Paese e dei cittadini,

riesce a risolverli attraverso l'interpretazione coerente, ma voi avete il dovere di eliminare problemi di costituzionalità, anche se sollevati solo come dubbio da una parte del Parlamento.

È un'ennesima normativa di urgenza che spoglia il Parlamento delle proprie prerogative, tra l'altro su materie per le quali non si riesce proprio a evincere quali siano i requisiti necessari di urgenza,

Tra l'altro, vediamo che all'interno del provvedimento si parla di disposizioni per l'efficienza del processo amministrativo. Ora, ricordiamo che qui non esistono nemmeno i requisiti e i riscontri fattuali, perché

il punto più dolente del decreto-legge è che si viene a discutere di una proposta di modifica

Si creano così delle situazioni evidenti di disparità di trattamento; sotto questo profilo, la norma non può non essere considerata viziata da profili di illegittimità costituzionale. Ma Ma ricordiamo qui, a tacer d'altro, il parere espresso dalla 1a Commissione permanente affari costituzionali del Senato; mi sento in obbligo, signori, proprio di richiamare testualmente tali parole, tra l'altro tenendo conto anche dello stesso profilo di valore espresso dalla 1a Commissione affari costituzionali qui al Senato, dove ci sono degli esimi ed illustri colleghi, che hanno titolo

1a Commissione, che ha rilevato evidentemente dei profili di illegittimità costituzionale. tematica che ritengo e riteniamo possa essere per certi versi ancor più grave, che dobbiamo assolutamente approfondire e che non possiamo far finta che non esista. La stessa 1a Commissione dice

in base ai quali la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente, all'interno del quale i magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni. Ciò che invece non avviene in questo disegno di legge di conversione del decreto-legge. Pertanto, questa palese e manifesta incostituzionalità, già rilevata, non può essere insignificante in questa sede e in questo dibattito; queste due norme non possono esistere nel nostro ordinamento e per questa ragione devono essere totalmente espunte. Noi, come Gruppo della Lega Nord, abbiamo proposto infatti emendamenti soppressivi proprio riguardo agli articoli 5 e 10. Dobbiamo veramente considerare che l'inserimento nell'ordinamento di una norma incostituzionale creerà sicuramente una problematica di tipo giudiziario, perché chi non usufruirà di questo trattamento avrà titolo e legittimazione per impugnare sicuramente la norma e rilevare il difetto di costituzionalità. Con ciò si dà vita a problematiche di difficile

che sono norme costituzionalmente illegittime che permettono al magistrato di Cassazione di permanere in servizio, creiamo una contraddizione in termini che al Paese non fa bene.

di una palese invasione e di una prepotenza esercitate continuamente dal Governo sul Parlamento. Per questa ragione, noi chiediamo che non si proceda all'esame del disegno di legge

posto che in esso sono contenute disposizioni ordinamentali alle quali difettano in maniera sostanziale le ragioni dell'urgenza dell'intervento in quanto si propongono di disciplinare una serie di

modificando la normativa relativa al mantenimento in servizio e al trasferimento dei magistrati, ai tirocini formativi e all'organizzazione del personale amministrativo. È di tutta evidenza, quindi, che non si tratta di necessità

del processo telematico amministrativo al fine di coordinare le regole tecniche con la normativa primaria per l'applicazione del PAT o di quella che istituisce, ad esempio, l'ufficio per il processo amministrativo, che sarebbe una nuova struttura di supporto nell'attività preliminare. È evidente a tutti che non ci troviamo di fronte a necessità urgenti e straordinarie, ma a modifiche che potevano essere introdotte attraverso un disegno di legge ordinario.

fosse finita la stagione delle norme *ad* *personam*!) è che qui ci troviamo di fronte a un decreto-legge palesemente *ad personam*.

in base al quale la legge è tenuta a regolare in maniera uguale situazioni uguali e utilizzare il principio di razionalità nel caso di situazioni diverse evitando discriminazioni arbitrarie e ingiustificate. Nello specifico l'articolo 5 assicura la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Corte di cassazione e la Procura generale della

il sistema di giustizia ordinaria e amministrativa) non è tale da giustificare tale deroga solo per alcune figure.

con la consapevolezza della certezza del diritto e quindi anche con la certezza del rispetto delle regole e con la differenza tra i buoni e i cattivi

sia ai giovani che agli anziani, che vengono mescolate, brillantemente e indifferentemente, con modifiche al sistema, che naturalmente vengono trattate in modo superficiale.

e gli altri magistrati, tutta la magistratura di merito, che conta un pochino meno. Quindi il grande rottamatore diventa il difensore della casta; non solo, il giovane rottamatore diventa il difensore degli anziani. Infatti, le questioni inerenti alla permanenza in servizio di questi magistrati potevano essere risolte in modo sicuramente molto più *smart* attraverso un sistema di reclutamento efficiente ed efficace; non è certamente togliendo ai giovani magistrati la possibilità di formarsi o riducendo il loro periodo di tirocinio che noi avremo una magistratura altrettanto preparata e messa rapidamente in servizio.

si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ma anche a quelli depositati alla medesima data, già depositati in precedenza,

che hanno presentato i loro ricorsi: ci sono quelli che avranno contezza di come verrà trattato il loro ricorso e quelli che "purtroppamente" avranno la sfortuna che non sia ancora stata decisa la data e quindi rientreranno in questa categoria "purtroppamente" e del tutto inconsapevolmente.

lasciassero il loro nome e cognome a tutti i cittadini che avranno legittimamente ragione per presentare le loro rimostranze: magari sono anche dei loro elettori, non si sa mai.

In ultimo vorrei far notare un altro aspetto paradossale, cioè che questo Parlamento (e segnatamente la Commissione giustizia) ha visto un *iter* di discussione del provvedimento in esame quanto mai arrogante e altrettanto incostituzionale:

di non poter fare alcun intervento, non perché non ci siano la volontà o l'intelligenza, ma semplicemente perché qualcuno ha deciso che della Costituzione se ne frega altamente: se ne frega del bicameralismo perfetto

spetterà ai Regolamenti regolare i diritti delle minoranze: se i Regolamenti saranno fatti da una maggioranza simile a quella che oggi gestisce il rapporto con le minoranze, direi che sarà molto difficile

signori del Governo, colleghi senatori, il provvedimento del quale stiamo discutendo evidentemente sta davvero molto a cuore all'Esecutivo, al punto da essere stato varato dal Consiglio dei ministri nel pieno dell'emergenza terremoto, quando non c'era il tempo per fissare la data del *referendum*, ma si è invece trovato il tempo per prorogare, per decreto-legge, il pensionamento del primo presidente della Corte di cassazione e di pochissimi altri magistrati apicali. tornerò sugli argomenti che evidenziano la dubbia compatibilità tra le misure al nostro esame e la Carta costituzionale: lo hanno fatto, meglio di quanto potrei fare, i colleghi che mi hanno preceduto. Vorrei invece osservare che questo atto, lungi dall'essere un fulmine a ciel sereno, si inscrive con straordinaria coerenza in una strategia di accentramento del potere che il Governo sta perseguendo perseguendo con pervicacia in ogni ambito. In altre stagioni, signora Presidente, per molto meno avremmo avuto il Paese in piazza, girotondi, allarmi

del "Governo più liberale del mondo" (spero che l'allegra brigata oltreoceano mi consenta la parafrasi da premio Oscar.

per potersi scegliere i dirigenti pubblici (a tal proposito lancio un allarme su come viene utilizzata la delega che il Governo ha in questa materia);

compie un salto di qualità. Con questo decreto-legge, nei fatti, il potere esecutivo sceglie i vertici dei principali uffici giudiziari italiani e i due membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura. Colleghi, non voglio essere ipocrita. L'attività di produzione delle leggi investe ogni ambito dell'ordinamento ed è dunque inevitabile che regoli anche la sfera di attribuzione di altri poteri dello Stato. Ma, tanto per cominciare, ciò dovrebbe avvenire nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento stesso. In secondo luogo, è disdicevole che ciò venga fatto

Soprattutto, quando un potere dello Stato interviene nei confronti di un altro potere dello Stato, è indispensabile porre attenzione a che tale intervento non dia adito nemmeno al minimo sospetto di strumentalità. Tante volte la politica ha preteso questa attenzione da parte dell'autorità giudiziaria: lo ha fatto anche il *premier* Renzi in quest'Aula. È dunque a dir poco sconcertante che oggi quello stesso Esecutivo dal quale tante volte abbiamo sentito scomodare Montesquieu, produca un atto così grave sotto il profilo dei rapporti tra i poteri dello Stato, così dirompente per gli equilibri all'interno dello stesso ordine giudiziario, così al di sotto di ogni sospetto. Presidente, vorrei continuare in questa linea di non ipocrisia. Il provvedimento che per decreto ha prorogato il trattenimento in servizio del primo presidente della Cassazione e di pochi altri eletti talmente poco dotato dei requisiti di necessità e urgenza che se ne parlava da mesi, come attesta un comunicato diramato già a giugno dai colleghi Giovanardi, Gasparri e Roccella - è stato magicamente licenziato dal Consiglio dei ministri dopo due episodi che in questa sede non intendo sottacere. Il decreto è stato varato dopo la sorprendente decisione del primo presidente della Corte di cassazione di non rimettere alle sezioni unite civili, come richiesto dalla procura generale, i ricorsi in materia di *stepchild adoption*, demandando la decisione ad una sezione della Suprema peraltro non presieduta dal magistrato che avrebbe avuto anzianità e titoli per farlo e che, proprio per questo, ha rassegnato le dimissioni dalla magistratura. È stato altresì dopo la decisione, ancor più sconcertante, di ammettere il *referendum* costituzionale senza provvedere a che il quesito da sottoporre agli elettori fosse conforme alle prescrizioni di legge. Tali prescrizioni sono chiarissime, signora Presidente. L'articolo 16 della legge n. 352 del 1970 opera infatti un'evidente distinzione tra leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale. In questo secondo caso, la norma impone che il quesito riguardi non l'oggetto della riforma, ma l'oggetto delle norme costituzionali sottoposte a modifica. A nessuno dei colleghi sfuggirà la differenza sostanziale. A nessuno sfuggirà quanto sia improprio e fuorviante richiamarsi alle richieste sottoscritte dai diversi promotori che, tenuti ad indicare burocraticamente la legge da sottoporre a *referendum*, lo hanno fatto mediante il titolo comparso in *Gazzetta Ufficiale*. A nessuno sfuggirà che se l'ordinamento detta regole vincolanti per la formulazione dei quesiti referendari, mentre nulla dice sui criteri di titolazione delle leggi, è evidente che il quesito non debba essere una mera trasposizione del titolo e la Cassazione non sia chiamata ad essere un semplice passacarte. A nessuno sfuggirà che evocare i precedenti del 2001 e del 2006 sia un chiaro *ballon d'essai*, se non un vero e proprio *boomerang*, dal momento che in entrambi i casi i titoli delle leggi di riforma si limitavano a perimetrare

legge Renzi-Boschi e come fa il quesito referendario che la Corte di cassazione ha così generosamente formulato. Presidente, colleghi, io non so se ricorrano i presupposti per - andreottianamente parlando - pensar male, anche se personalmente mi sono fatto un'idea abbastanza chiara di questa vicenda. Certamente i presupposti di costituzionalità non ci sono. E un'altra cosa è certa. Sapevamo già, al di là delle ambizioni tipiche del suo carattere, di non essere governati da un personaggio

E questo, in un contesto di occupazione del potere sempre più spregiudicata e soffocante, è qualcosa che dovrebbe preoccupare tutti, non soltanto noi dell'opposizione.

sono completamente incostituzionali, al punto che il sottosegretario Chiavaroli si sarebbe fatta carico di trasferire al ministro Boschi l'esigenza di stralciare o modificare i due articoli in oggetto.

dico che questo testo deve essere fermato attraverso la questione pregiudiziale? Perché tutto quello che noi stiamo facendo in questo periodo è teso e finalizzato solo allo svolgimento e all'esito favorevole del *referendum*. Il Senato non fa nulla di divisivo, come ho già detto. Si approva una legge di stabilità perché è obbligatoria, distribuendo prebende a tutti pur di raccogliere consenso, già sapendo che arriverà la lettera di richiamo dell'Europa, il cui effetto si produrrà a babbo morto, cioè dopo il voto del 4 Ma per potervi arrivare è necessario che il *referendum* si possa svolgere, ovvero che vi sia stato il passaggio in Cassazione, dal Presidente della Repubblica e l'esame da parte dei ricorrenti presso la giustizia amministrativa. Casualmente, l'articolo 5 e l'articolo 10 contengono i posticipi dei pensionamenti dei vertici apicali della Cassazione e del Consiglio di Stato. qualche dubbio sulla coincidenza di questi passaggi francamente ce l'ho. Chi ha dichiarato, come ricordava prima il collega, l'ammissibilità dei quesiti referendari in Cassazione? in Cassazione? Proprio quelli che usufruirebbero del posticipo del pensionamento! A chi oggi è rivolta la domanda se il quesito sia o no ammissibile? Alla giustizia amministrativa, cioè al Tar, e dopo, eventualmente, al Consiglio di Stato. Tale quesito era, ed è, completamente inammissibile. Non tanto perché fuorvia la volontà dell'elettore, ma perché, *per tabulas*, il Senato, come era e come sarà, è un organo costituzionale obbligatorio. Quindi, la legge elettorale che andrà a eleggerlo è una legge costituzionalmente obbligatoria. *Per tabulas*, come ormai sanno anche gli asini,

ha scritto che il consigliere regionale voterà per una lista di consiglieri e di sindaci. Ma si dice anche che la lista che prenderà più voti, cioè il vincente, ha il diritto di optare nella scelta tra consigliere e sindaco. Peccato ci si sia dimenticati del fatto che dieci Regioni hanno solo due senatori e che in alcune (e abbiamo già fatto le simulazioni) tutti e due gli esponenti andranno alla maggioranza. Se la maggioranza che ha vinto opta per il sindaco, in quella Regione si avranno due consiglieri e non si avrà il sindaco. Quindi, settantacinque consiglieri e venti sindaci:

è di consiglieri o di sindaci o se debbano essere due. Ma sono ancor più perplesso rispetto al fatto che qualcuno proponga di fare in fretta una legge a regime. Peggio mi sento, perché, in base all'articolo 2, non è scrivibile una legge elettorale per l'elezione del Senato. Non si può infatti scrivere che bisogna eleggerlo con il sistema proporzionale e, quindi, con l'attribuzione dei seggi in funzione dei voti espressi (cioè la proporzionalità) e della composizione del Consiglio. La proporzionalità è una cosa, la composizione del Consiglio è un'altra in quanto viene da un sistema maggioritario perché, tranne una Regione, tutte le altre hanno una legge elettorale maggioritaria.

in dieci Regioni ci saranno solo due senatori. Qualcuno mi vuole spiegare come fa a essere proporzionale l'attribuzione di quei due seggi

per volerci sciacquare la bocca con qualcosa che passa sempre, si promuove l'equilibrio di genere. Allora, mi spiegate quei due senatori come devono essere fatti?

In primo luogo si dice che il diritto di difesa, ma soprattutto il diritto al contraddittorio, sarebbe offeso dalle disposizioni delle quali ci stiamo occupando e, segnatamente, dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge. Intanto, mi permetto di ricordare che il contraddittorio ha diverse facce nel nostro sistema costituzionale. È un metodo di formazione della prova e, se intendiamo per contraddittorio il metodo di formazione della prova, dobbiamo convenire che, dinanzi alla Corte di cassazione e nelle giurisdizioni di legittimità, la prova certamente non si forma. Quello è un giudizio che implica la già avvenuta formazione della prova nei gradi di merito del giudizio. Certo, non nego che la trattazione in pubblica udienza determini l'espansione di una forma diversa di contraddittorio, il cosiddetto contraddittorio consistente nel conflitto tra le parti che, in un certo senso, manifestano le loro diverse opinioni in un'udienza pubblica. Questa possibilità di espansione di un contraddittorio, che può essere anche cartolare perché nessuna norma vieta che il contraddittorio sia tale, è recuperata nei casi di eccezionale o di particolare rilevanza delle questioni poste. Infatti, in presenza della straordinaria o eccezionale rilevanza delle questioni, il presidente può disporre che il ricorso sia portato nell'udienza pubblica. Quindi, abbiamo l'affermazione di ordine generale che non confligge né con l'articolo 24 e nemmeno con l'articolo 111 della nostra Costituzione, secondo il quale il contraddittorio può essere anche di natura cartolare. Il conflitto tra le diverse posizioni processuali si può risolvere anche attraverso scritti che vengono depositati dalle parti in un contesto normativo che prevede, pur sempre, la possibilità, in presenza di situazioni che lo meritino, di portare le questioni in udienza pubblica. Passando alla questione di costituzionalità successiva, che riguarderebbe la violazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione e, quindi, gli articoli 5 e 10 del decreto-legge,

3. Infatti, non dobbiamo dimenticare come, tutte le volte in cui si discute di pretese violazioni del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza, le questioni vadano in un certo senso concretizzate, cioè vadano esaminate nel loro contesto. Qui abbiamo un presupposto sul quale tornerò successivamente, con riferimento all'ulteriore questione sollevata, ossia la pretesa violazione dei requisiti di necessità e d'urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione per dire che alla base del decreto-legge vi sono non soltanto l'urgenza e la necessità (che ne legittimano l'adozione, appunto, sul versante dell'articolo 77), ma anche la straordinarietà delle questioni trattate attraverso l'adozione di questo decreto-legge. È attraverso questo prisma della straordinarietà delle questioni, della loro importanza, dell'eccezionalità e della crisi

presentato secondo il versante che più aggrada coloro i quali sostengono una certa tesi, e in quel separato contesto acquisiscono una forza di persuasione che in realtà non hanno. È l'arte del convincere e in un certo senso il sofisma che si presenta a determinare una certa credibilità, soltanto apparente, della questione. Il punto di partenza, anche sul versante dell'uguaglianza e della ragionevolezza, non può non essere costituito dalla necessità di affrontare un'emergenza che si caratterizza per un numero di ricorsi straordinariamente elevato: se abbiamo 106.000 ricorsi pendenti, che sono esattamente il doppio del numero dei ricorsi pendenti solo dieci anni fa, dobbiamo inevitabilmente comprendere che occorre adottare misure che, seppure nel rispetto dei principi costituzionali, rispondano a queste esigenze di straordinaria eccezionalità. Questo è un punto di partenza nella valutazione dei requisiti di costituzionalità, *ex* articolo 3, congiuntamente anche al presupposto dell'articolo 3:

la Corte di cassazione è in sé elemento giustificativo di disposizioni che riguardano direttamente la Corte di cassazione. Vedano, signori senatori e signore senatrici, come la questione in un certo senso finisce per dare ragionevolezza, al contrario di quello che si pretende di fare, a questo intervento legislativo, nella misura in cui, premessa la straordinarietà della situazione nella quale versa la Corte di cassazione, premessa appunto la necessità di disporre in maniera differenziata situazioni che sono differenziate, si dispongano norme introduttive di un trattamento separato, data l'emergenza, per i ricorsi di Cassazione, e si intenda accompagnare l'entrata in vigore di disposizioni eccezionali, attraverso la permanenza degli uffici di vertice della Corte di cassazione, che al contrario sarebbero stati contestualmente decapitati. Quindi, c'è una ragionevolezza di fondo in un intervento che, per l'appunto, mira a risolvere un problema specifico attraverso disposizioni specialmente dettate per questa situazione particolare e che includono, all'interno di tale situazione, una proroga del pensionamento degli uffici di vertice della Corte di cassazione, e poi inevitabilmente delle altre magistrature superiori. Se questo non fosse stato fatto, si sarebbe rinvenuta una disparità di trattamento all'interno delle magistrature superiori, nel senso che si sarebbe regolata diversamente una magistratura superiore rispetto ad un'altra; superiore rispetto ad un'altra; ma nessuno può ragionevolmente dire che un ufficio direttivo di una Corte d'appello costituisca una situazione identica un ufficio direttivo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. Per quanto riguarda gli articoli 104 e 107 della Costituzione, le relative obiezioni in un certo senso confluiscono nella critica di cui all'articolo 3; poi, certo, i magistrati si possono distinguere solo per funzioni, ma qui il principio non è assolutamente vietato per l'ovvia ragione che si stabilisce una deroga in materia di pensionamento in virtù, per l'appunto, delle situazioni alle quali inizialmente mi riferivo. riferimento all'articolo 77, laddove si dice che mancherebbero i requisiti di necessità e urgenza, per ricordare come proprio i dati statistici, e cioè la particolare situazione nella quale la Corte di cassazione si trova, costituiscono testimonianza evidente di una situazione di assoluta urgenza. Per tutte queste ragioni mi permetto di ritenere che le questioni di costituzionalità proposte

e di distinguere la posizione che io rappresento questa mattina - che peraltro non è isolata - anche dalle argomentazioni svolte dal collega D'Ascola per ultimo. Intanto desidero ringraziare il relatore per la sua relazione trasparente: il relatore, nel riferire sul provvedimento, non ha nascosto alcuno dei problemi sul tappeto e, anzi,

guardate rigorosamente con i criteri classici dell'omogeneità, potrebbero sicuramente far protendere la bilancia in un altro verso. Noi pensiamo, però, che l'omogeneità sia salvaguardata dall'obiettivo

al dovere di testimonianza che hanno i senatori della Repubblica e i parlamentari tutti rispetto ai provvedimenti di rilevanza particolare; e questo è un provvedimento che ha una rilevanza particolare e, su alcuni punti, sicuramente non positiva. Siamo consapevoli peraltro che la 1ª Commissione omologa della Camera dei deputati ha fatto ragionamenti di tipo completamente diverso.

ha una forma di rispetto nei confronti della prima. Ma ora, se volessi essere leggermente polemica (e, visto che stiamo discutendo dell'Italicum in tutti i luoghi, lo voglio essere dichiaratamente), dovrei dire che quanto è successo alla Camera non mi fa ben non mi fa ben sperare per il futuro perché, se quando le maggioranze sono blindate non si vedono neanche le cose per le quali non bisogna certo inforcare un paio di occhiali per vederle, ciò non depone bene per il futuro. Ritorno alle motivazioni.

tutto inappropriata, ma anche gratuita, norme assolutamente discriminatorie. Oggi lo diciamo nell'Assemblea del Senato e lo dico anche a nome di un gruppo di senatori che la pensano come me all'interno del PD sono molti di più a pensarla così, molti di più di quelli che lo dichiarano). In realtà non siamo i primi a dirlo. L'ha detto l'Associazione nazionale magistrati e l'ha detto il Consiglio superiore della magistratura, con un provvedimento (naturalmente riferito alla giustizia amministrativa e quindi al presidente e al procuratore generale della Corte di cassazione) molto analitico e molto motivato, che portava il Parlamento davanti a un bivio: cassare cassare i due articoli o modificarli. Non ci sarebbe stato niente di scandaloso ad emendare questi articoli in maniera non discriminatoria, cioè disciplinando

allora non si vede come, nascondendosi dietro a un apparato organizzativo e quindi dietro ad un ufficio, si possa consentire ad alcuni magistrati una proroga, mentre si tralasciano e si discriminano tutti gli altri magistrati, con conseguenze anche personali che probabilmente porteranno La collega De Petris, ma anche qualcun altro, ha poi fatto riferimento ad un altro articolo, al quale vorrei fare riferimento anch'io in questa mia breve discussione, cioè l'articolo 7.

avere la velina ai singoli parlamentari per introdurre per via parlamentare quello che non riescono ad introdurre per via governativa. a chi è potuto venire in mente? Al collega Ermini della Camera (responsabile giustizia del PD) come poteva venir in mente di inventarsi che l'ufficio di presidenza, in determinate condizioni, ha bisogno di due elementi suppletivi individuabili in maniera così analitica? Dico questo perché, tra l'altro, questo articolo non poteva sfuggire; infatti non è sfuggito a me, alla collega De Petris e alla Commissione (che però non si è pronunciata, perché era fuori dal decreto-legge). Non poteva sfuggire, perché ha suscitato le proteste dei magistrati del TAR, che si sono visti messi in un angolo e che conteranno molto

autonoma e indipendente (e in questo momento la tuteliamo o la dovremmo tutelare anche dalle discriminazioni), ma abbiamo bisogno anche di un potere legislativo indipendente, perché non è possibile che singoli magistrati dettino l'agenda politica del nostro Paese, né quando fanno introdurre né quando fanno introdurre norme che li riguardano personalmente, né quando fanno introdurre norme con modifiche subdole, che non si capisce con quale ragionamento vengano introdotte e che favoriscono alcuni a discapito di altri o alcune categorie a discapito di altre. Dunque, alla fine di questo discorso ci sono emendamenti che, se dovessero

Se guardate i giornali di questa mattina, vedrete che parlano, personalizzandolo, di un decreto-legge che è stato pensato - ahimè - per premiare alcuni magistrati (manca solo la foto di questi magistrati). Poi si è usato un *escamotage* per dire che non si tratta solo della Cassazione, ma anche del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. A me risulta che non ci sia alcun magistrato della Corte dei conti e del Consiglio di Stato che possa beneficiare di questa proroga *ad personam*.

era obbligatorio che i ricorsi andassero alla sezioni unite della Cassazione. Invece no. Il presidente Canzio ha scritto a noi parlamentari che, anche se la legge prevede che se ne occupino le sezioni unite, lui, seguendo la prassi, li ha affidati alla prima sezione, che, come ha detto

discusso - non si sa perché - dalla sesta sezione, e solo a seguito della nostra protesta la sesta sezione si è spogliata di questo compito rimandandolo alla prima sezione. E noi ribadiamo la richiesta, come la legge prevede, di dare alle sezioni unite la funzione che esse hanno nel nostro ordinamento:

essendo i contratti di convivenza uomo-donna parificabili alle unioni civili tra uomo-uomo o donna-donna, ed essendo questi paragonabili al matrimonio, d'ora in poi basta un contratto di convivenza e il clandestino che ha commesso reati nel nostro Paese non può più essere espulso.

Veniamo al dunque. Sarebbero questi gli atteggiamenti per cui il primo presidente viene premiato con una proroga di un anno, lui e alcuni membri della Cassazione? Il senatore Quagliariello ha anche sottolineato il quesito referendario, che ha avuto un certo tipo di interpretazione. Ma voi pensate che nel Paese, nel Consiglio superiore della magistratura e a livello dell'Associazione nazionale magistrati (che ha criticato aspramente questi provvedimenti), nessuno si sia accorto nessuno si sia accorto che addirittura vengono imbrogliate le carte non soltanto con l'occupazione delle televisioni e dei giornali, magari con un accordo tra il Ministero della sanità e qualche potente imprenditore della sanità per far fuori la sera, alle ore 20, il direttore di un giornale per farla passare, dalla mattina alla sera, dal «no» al «sì» rispetto Non solo si occupano queste posizioni del giornalismo o si riempiono tutti gli enti di Stato con persone che arrivano dal Granducato di Toscana o dalle sue vicinanze, ma addirittura si adottano decreti-legge per "premiare" persone

che entra nel merito e ridisegna le funzioni della Corte di cassazione. Eppure ciò viene fatto con disinvoltura, si stracciano le regole costituzionali in maniera assolutamente disinvolta e si ignorano le sentenze della Corte costituzionale. A meno che non si prefiguri una realtà istituzionale in cui la Corte costituzionale

è bene chiamarle per nome e cognome e stabilire le responsabilità. Poiché il tempo è galantuomo, ci sarà il momento in cui queste cose verranno rivalutate e riviste, spero anche a livello istituzionale, e chi compie queste forzature incredibili ne pagherà le conseguenze, davanti alla storia, davanti al Paese e spero anche a livello elettorale.

prossimità. Su questo gradirei avere il parere e una presa di posizione da parte del Presidente del Senato, in considerazione del fatto che ciò potrebbe costituire un precedente grave, per i lavori e per lo stesso principio di funzionamento democratico dell'istituzione.

Credo che un titolo più corrispondente al contenuto principale del provvedimento avrebbe potuto essere: «Misure urgenti per il mantenimento in servizio di sei o sette figure apicali della Corte di Cassazione»

che ha anticipato di cinque anni la data di pensionamento dei magistrati, senza prevedere i corrispondenti concorsi per la loro sostituzione, infischiandosi delle prevedibili conseguenze sul piano del corretto funzionamento della giustizia». Questo sarebbe stato forse il titolo più adatto, più corretto e più legittimo per il disegno di legge

perché in un momento in cui a tutto il Paese viene chiesto di andare in pensione un po' dopo, di spostare in là l'asticella,

anche perché la richiesta di considerare dei periodi transitori era stata avanzata dal Consiglio superiore della magistratura, dagli stessi magistrati, dalle forze politiche, ma ovviamente tutte queste istanze sono state Siamo quindi giunti alla terza proroga. Rimane un interrogativo: perché questa proroga, a parità di condizioni, non è stata prevista per tutti i

Perché è stato introdotto questo precedente, questa discriminazione tra giudici di legittimità e di merito? Signor Presidente, si sta introducendo una disparità di trattamento incredibile che innescherà inevitabilmente innumerevoli ricorsi da parte degli stessi magistrati. La dichiarazione di incostituzionalità del provvedimento in esame, quantomeno perché contrario agli articoli 3 e 107 della Costituzione, è certa: è solo una questione di tempo. Per fortuna, grazie alla Costituzione, che è ancora vigente nel nostro Paese nonostante ci siano reiterati tentativi di stravolgerla, i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge e i magistrati si distinguono tra loro soltanto per la diversità di funzioni. nel 2014 è stata lanciata dal *Premier* la cosiddetta parabola del ricambio generazionale in magistratura, poi però non si è provveduto a fare i concorsi, a fare i concorsi, a coprire i posti che sono stati lasciati vacanti a causa dei prepensionamenti, non si è provveduto con le assunzioni e con le assegnazioni e poi ci si chiede perché in Italia la giustizia non funzioni.

non è altro che l'ennesima riprova. Anche l'Associazione nazionale magistrati ha dichiarato che il testo presenta profili di incostituzionalità ed è in contrasto con il diritto comunitario.

mi rivolgo, attraverso questa Assemblea, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e anche al Presidente del Senato, che è persona che il diritto lo conosce e lo pratica ancora più di noi parlamentari che pure, facendo le leggi, qualcosa abbiamo appreso. Questo provvedimento, infatti, sul quale il Governo si accinge a porre la fiducia, è di una tale incostituzionalità che non ci sarebbe bisogno della verifica che su un decreto-legge la Presidenza della Repubblica deve comunque fare nel momento in cui lo firma e ne autorizza l'avvio dell'*iter* parlamentare. Poi, dovrà essere promulgata la legge di conversione; quindi, un decreto-legge passa due volte al vaglio della suprema magistratura della Repubblica: sia quando lo

non voglio farli; credo siano 13 le persone - stanno tutte in Cassazione - beneficiarie di questa norma. Anche sulla tecnicalità del problema delle proroghe, o dei vuoti che si creano per altri provvedimenti, non aggiungo nulla a ciò che altri colleghi esperti assai

Abbiamo visto l'auto-ostruzionismo della maggioranza, perché il diavolo fa le pentole ma non i coperchi: arruolano i senatori transfughi per reggere il Governo ma poi il transfuga, casomai sul processo penale, non è d'accordo - in un barlume di lucidità - sulla prescrizione che arriva fino a trentatré anni e allora il Governo non ha i numeri

per legge a sezioni unite e non decide; forse ha anche poco coraggio, perché l'altro giorno siamo andati democraticamente davanti alla Cassazione a esporre uno striscione: era attesa una decisione della sesta sezione, è stata trasferita alla prima. Non si è ancora deciso, ma su materie come le adozioni, che sono delicatissime, dovrebbero pronunciarsi le sezioni unite. Si preoccupano di avere la pensione *ad personam* prorogata e non si preoccupano di applicare la legge in modo corretto sul tema delle adozioni! Hanno fatto quello che hanno fatto l'altro giorno, applicando in Cassazione

Non farò i nomi del procuratore della Cassazione generale, dei presidenti di sezione, dell'avvocato generale presso la Cassazione: basta andarli a vedere su

metterci la fiducia è banditismo raddoppiato e lo sanno anche i colleghi che voteranno la fiducia. Ho sentito qualche eco e ho letto i pareri della Commissione giustizia: è uno schifo!

Presidente, dirò cosa penso di questo provvedimento in sede di dichiarazione di voto. Non volevo però perdere anche questa occasione per evitare che il Parlamento prenda una deriva sulla quale francamente non si può continuare a soprassedere. Presidente Calderoli, le chiedo un attimo di attenzione, perché siccome so che il presidente del Senato

A me viene in mente una cosa molto semplice. Pensando a questo provvedimento, mi ricordo una frase di un valoroso polemista italiano, Ennio Flaiano, il quale si perché si continua a spostare sempre più in là la soglia del ridicolo? Questo è il pensiero che mi fa venire in mente questo provvedimento e le chiedo di fare attenzione con me su alcune questioni di metodo, perché molto spesso il metodo diventa sostanza in questo Parlamento. Non possiamo essere convocati dalla Commissione giustizia il lunedì sera per una seduta notturna, paventando un problema di urgenza, e trovarci il giorno dopo, cioè ieri, con una maggioranza che ci impone l'inversione dell'ordine del giorno e discutere di altro. Sta succedendo veramente qualcosa di inammissibile. Gli spazi delle opposizioni vengono completamente calpestati. Chiedo allora a lei, in funzione di Presidente in questo momento credo che anche altri se ne dovrebbero interessare - cosa sta succedendo in questo Parlamento rispetto, ad esempio, alla decretazione d'urgenza. Se i moniti del recente passato continuano ad avere diritto di cittadinanza in queste Aule parlamentari, possibile che ci sono Presidenti della Repubblica che viaggiano a senso alternato? O devo pensare che tutto sta nella logica che ha animato, ad esempio, l'intervento che ha fatto prima la senatrice Lo dove c'è tutto e il contrario di tutto, dove praticamente si recitano dieci parti a soggetto in scena? Siamo nella completa inconsistenza completa inconsistenza dei lavori dell'Aula, nella completa inconsistenza dei lavori parlamentari su provvedimenti di cui parlerò poi in dichiarazione di voto e che segnalerò

ero in missione venivo bombardata sul mio cellulare di messaggi della Commissione giustizia, che in modo disorganizzato e frenetico

che io pure avevo presentato e che, legittimamente, avevo anche il desiderio di poter votare, oltre che di potermi esprimere sul loro contenuto. È evidente che l'organizzazione di questa riunione della Commissione in seduta notturna è avvenuta con la piena responsabilità e consapevolezza di una maggioranza che si è attrezzata, che si è organizzata per le sostituzioni e che ha

votare. Questo è il segno più evidente, tangibile e concreto, di un Governo che ha occupato di fatto il ruolo dei parlamentari, che comunque sono stati eletti e che, comunque, hanno il diritto e il dovere di rendere conto alle persone che li hanno eletti. Questo nella più completa indifferenza dei colleghi senatori,

comunque, non interessa a coloro che hanno la pretesa di guidare questo Paese. Non parliamo poi delle questioni di costituzionalità e incostituzionalità, già ampiamente trattate e che restituiscono il quadro di operazioni fatte nel più completo spregio della Carta costituzionale. Spregio dei meccanismi parlamentari, spregio della rappresentanza, spregio della Carta costituzionale: qualcuno, qui, dovrebbe veramente vergognarsi. Per quanto riguarda il merito di questo provvedimento, ancora una volta ci troviamo davanti un decreto-legge riguardante la giustizia. Mai abbastanza si è osservato che la giustizia avrebbe bisogno di provvedimenti che vadano prima di tutto a toccare i veri punti dell'efficienza e del funzionamento della macchina; problemi che vengono sempre costantemente risolti per *spot*. c'è anche l'aggravante di un trattamento dispari e della creazione, di fatto, di una piccola casta. Quindi, aggiungiamo anche la decretazione *ad personam*. Ma io vorrei fare anche una riflessione su qualcos'altro, cioè sul concetto di legalità. Nel mondo esterno a questa Camera, presa amabilmente a calci nel sedere,

protocolli. Ebbene, vorrei far notare che, comunque, la legalità e il principio del rispetto delle regole non sono dichiarazioni e petizioni di principio, ma ma comportamenti rispetto ai quali il modello è fondamentale, perché diventa un modello educativo. Ci troviamo allora davanti a un Governo che esprime un pessimo modello quanto a rispetto delle regole, perché delle regole se ne infischia altamente. Non è certamente esemplare. Ci troviamo davanti a una serie di provvedimenti che si accavallano e che sono uno la negazione dell'altro.

siamo impossibilitati ad affrontare un provvedimento che è pronto; mi riferisco alla riforma del processo penale, rispetto alla quale ci sarebbe molto da dire, ma che comunque è qui: è stato votato in Commissione, è disponibile per l'Assemblea, ma non lo possiamo affrontare. Giace anche il provvedimento che riguarda la riforma del processo civile. Pur essendo provvedimenti disomogenei, sono tuttavia provvedimenti che hanno seguito un *iter* parlamentare e che avrebbero l'ambizione di affrontare in modo più organico sia il fronte della giustizia penale, che quello della giustizia civile. Questi provvedimenti, che comunque giacciono, sono in netto contrasto - e mi metto avanti sui lavori - con altri provvedimenti. altri provvedimenti. Abbiamo avuto già qualche anticipazione e sappiamo quali temi conterrà la prossima legge di stabilità. Penso, per esempio, alla rottamazione delle cartelle

quel dovuto che viene pagato, ma che non è stato pagato a tempo debito, si è tradotto nella fatica degli insegnanti, per esempio, che si sono ritrovati ad avere in classe trenta studenti. Bisogna tagliare sulle spese della scuola perché il dovuto non viene pagato

per il concetto di rispetto della legalità. A suo tempo è stata resa più appetibile con l'istituzione e immediata depenalizzazione dell'autoriciclaggio. Qui invece, siccome non si può più istituire per depenalizzare l'autoriciclaggio, si fa la *voluntary disclosure* addirittura sul contante, il che significa che si fa una brillante operazione per allestire una lavatrice di denaro di qualunque provenienza.

per poter guidare questo Paese fuori da una crisi economica che, prima di tutto, ha messo in crisi il valore stesso della democrazia.

di un decreto-legge che è stato discusso ampiamente in Commissione. Lo stesso relatore ha dato atto delle sedute che sono state ampiamente dedicate all'approfondimento dei

che questo decreto-legge non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma fa parte di una strategia più globale e sistematica

la riforma della giustizia non è più un motivo di scontro ideologico, ma diventa finalmente un motivo di elaborazione di testi e poi di approvazione di leggi. Il dibattito c'è, ci sono conflitti, divergenze e convergenze, ma non c'è lo stesso clima di qualche anno fa.

punti, qualificati dalla necessità e dall'urgenza, che sono stati tenuti in piedi in questi mesi di legislazione. Ricordo a tutti i colleghi che è in corso di approvazione (perché già un ramo del Parlamento, il Senato, l'ha approvata) la riforma della giustizia civile;

non siamo ai suoi tempi, quei tempi che fecero molto male al sistema Paese, ma siamo in un'altra fase. Ecco perché respingiamo al mittente tutte quelle

Insomma, cari colleghi, ci troviamo di fronte a un decreto‑legge il cui chiaro intento è intervenire su una situazione di smaltimento dell'arretrato che riguarda in modo particolare la Corte di cassazione.

che la Corte di cassazione possa finalmente aggredire l'arretrato, soprattutto quello civile, e dare una risposta adeguata. Il Presidente della Commissione lo ha ricordato: ci troviamo, dagli inizi degli anni Novanta, di fronte a un arretrato pendente micidiale.

ci siamo aggirati sempre intorno a questa cifra e ci troviamo oggi, al 30 giugno del 2016, intorno ai 106.000 arretrati. Ecco perché, cari colleghi, questo è un dato certo, inoppugnabile e oggettivo con cui dobbiamo fare i conti. Si dà una prima, parziale, limitata ma interessante risposta. Anche questa è una discussione che avveniva da anni nella quale ci si chiedeva se utilizzare quel gruppo qualificato di magistrati di merito che lavorano al delicato compito del massimario, naturalmente non in modo occasionale ma rispettando le tabelle di organizzazione della Corte e le stesse esigenze dell'ufficio del massimario.

In sostanza si generalizza l'uso della trattazione in camera di consiglio nei procedimenti civili che si svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte e si modifica anche la procedura del cosiddetto filtro in Cassazione. Anche questa è una norma discussa, elaborata e contenuta, seppure in forma di delega, nella legge di riforma del processo civile già approvato dalla Camera, come ho detto prima, e in valutazione qui da noi al Senato.

riforma i ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione - va da sé - e quelli per i quali non è stata ancora fissata l'udienza o adunanza in camera di consiglio.

presso la Corte di cassazione, stabilendo che l'attività di formazione degli ammessi allo *stage* sia condotta in collaborazione con il Consiglio nazionale forense, nonché con le scuole di specializzazione per le professioni legali. citato anche questa ulteriore norma per far capire che si sta intervenendo in modo sistematico per affrontare il tema dell'arretrato in sede di Cassazione. E ancora, cari colleghi, si allarga lo spettro dell'intervento e si fanno anche degli inserimenti, molto interessanti e importanti, nel campo più generale della giustizia. Sempre all'articolo 2, commi 2 e 5, si interviene sulla disciplina del concorso per magistrato ordinario, consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero dei posti in bando al concorso in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici e si riduce, in via eccezionale, da diciotto a dodici mesi la durata del tirocinio dei magistrati che saranno nominati a seguito dei concorsi già banditi nel 2014 e nel 2015 per consentire alle nuove leve di svolgere quanto prima la funzione giudiziaria. Devo dire che anche in questo caso si è intervenuti in modo intelligente, senza lasciare scoperta questa attività preziosa

poter così vincere un difficilissimo e selettivo concorso) e si è voluta, invece, rafforzare la parte che li colloca già presso gli uffici giudiziari.

di trattenere in servizio fino al 31 dicembre 2017 coloro che abbiano compiuto il 72o anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la data predetta e il 30 dicembre 2017. Si tratta si possono individuare diverse soluzioni, tutte legittime, ma nessuno può avanzarne una e dire che le altre sono norme *ad personam* o addirittura sono viziate da incostituzionalità. Il dibattito è sempre aperto. Il Governo ha scelto un percorso e penso che questo possa essere valutato nella sua consistenza e nel merito. Penso anche che questa scelta possa essere sostenuta. Ecco perché, cari colleghi, anche in tutte le altre norme presenti in questo decreto-legge, c'è un ulteriore tentativo di fare in modo che il nostro sistema giustizia sia riformato, innovato e migliorato.

Presidente, vorrei esprimere un generale apprezzamento per i contenuti di questo decreto-legge, poiché il provvedimento è finalizzato a raggiungere un'efficace composizione tra le diverse esigenze che devono essere soddisfatte nell'amministrazione della giustizia, all'urgenza di assicurare celerità e sburocratizzazione dei procedimenti, alla necessità di assicurare condizioni di lavoro che favoriscano la professionalità e l'efficienza dei magistrati. Intendo quindi fare riferimento ad alcuni passaggi significativi del disegno di legge: *in primis* la previsione dell'articolo 1, in forza della quale i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo possono essere impiegati eccezionalmente per comporre i collegi giudicanti, tanto civili quanto penali, della Corte di cassazione, con la giusta finalità di rafforzare i presidi organizzativi necessari ad un più rapido smaltimento dell'arretrato. Sempre trattando questo argomento, è apprezzabile l'intervento della Camera in prima lettura, che ha limitato l'applicazione della disposizione ai soli magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità e ponendo un limite triennale non rinnovabile. All'articolo 2 si prevedono misure per migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari: per coprire i vuoti di organico della magistratura ordinaria, si aumenterà sino a un decimo il numero dei posti disponibili tra quelli messi a concorso nel biennio 2014-2015; inoltre, sarà possibile ottenere una più rapida copertura dei posti vacanti nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado attraverso la riduzione del tirocinio, da diciotto a dodici mesi, dei magistrati dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015. Inoltre, per quanto riguarda la normativa dell'articolo 3, vorrei sottolineare come essa riguardi esclusivamente il periodo di legittimazione un magistrato può fare domanda di trasferimento ad altro incarico o ad altra funzione. L'allungamento a quattro anni è dettato dalla considerazione, peraltro facilmente condivisibile, che il termine triennale non sia pienamente sufficiente affinché il magistrato possa dare un contributo effettivo al pieno assolvimento degli incarichi assegnati: nel momento in cui si entra in un sistema, infatti, dobbiamo garantire un orizzonte temporale che metta il magistrato nelle condizioni di svolgere quella funzione con la necessaria progettualità delle scelte dell'ufficio e con la più alta stabilità della posizione, prerequisito per il pieno manifestarsi di professionalità e capacità. Ritengo quindi vada nella direzione giusta anche la norma dell'articolo 4, finalizzata a sfruttare tutte le risorse umane disponibili all'interno degli organici: si stabilisce, infatti, che il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e il personale assegnato agli uffici di sorveglianza non possa essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza. Parallelamente e coerentemente, fino al 31 dicembre 2019 il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia non potrà essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni. L'intervento degli articoli 5 e 10 del decreto-legge, lungi dal rappresentare violazioni dei principi relativi all'uguaglianza e alla parità di trattamento, tantomeno ingerenze nelle competenze di un ordine autonomo ed indipendente come la magistratura,

Il Capo II del decreto-legge è dedicato al processo amministrativo telematico. Gli articoli in questione recano importanti previsioni finalizzate a consentire l'entrata in funzione del processo amministrativo telematico, dettando precise norme di coordinamento ed adeguamento della disciplina a principi di buon senso, funzionalità e semplicità degli adempimenti. Nello specifico, i nuovi meccanismi procedimentali basati sulla tecnologia, il cui avvio è già previsto per il 1° gennaio 2017, saranno promossi semplificandone l'operatività, attraverso l'introduzione di misure atte ad armonizzare gli strumenti del processo amministrativo telematico con il codice dell'amministrazione digitale. Mi riferisco in particolar modo al domicilio digitale e all'estensione agli avvocati difensori della attestazione dell'efficacia probatoria delle copia per immagine di documenti cartacei. Allo stesso obiettivo tendono le misure finalizzate a estendere l'utilizzo delle modalità di deposito degli atti anche per i soggetti non dotati di posta elettronica certificata.

certificata. Per concludere, colleghi, questo è un provvedimento di urgenza che, dopo essere stato anche debitamente integrato dal Parlamento, fornisce degli strumenti rapidi, concreti ed efficaci per continuare ad aggredire, al di là delle solite e sterili critiche preconcette, i mali cronici che affliggono il settore della giustizia del nostro Paese.

lì) i procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione alle sezioni civili, di cui

ha indotto il primo presidente della Corte di cassazione ad applicare alle sezioni civili anche i giudici applicati al penale, i quali però sono presenti nelle varie commissioni tributarie, proprio per smaltire quei 45.000 procedimenti pendenti. Si una situazione di straordinaria eccezionalità. muovere rilievi, anche da colleghi autorevolissimi e da giuristi autorevoli, in tema di incostituzionalità del decreto-legge.

«Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione». ragionevole durata del processo. Non è forse questo, colleghi, un principio affermato nell'articolo 111 della Costituzione? E, se si adotta un provvedimento che va nella direzione di vedere applicato un principio della Costituzione, come si può giammai parlare di provvedimento incostituzionale? Il ragionamento del presidente D'Ascola per la verità è ineccepibile: la violazione della norma in rapporto all'articolo 3 della Costituzione (quindi al tema dell'uguaglianza) deve presupporre che le due condizioni siano identiche. L'idea di valutare le medesime difficoltà anche presso altri uffici giudiziari idea ovviamente interessante, proprio per evidenziare la disparità di trattamento venne in Commissione giustizia a un raffinato giurista, il presidente Nitto Palma, il quale chiese al Sottosegretario di conoscere i dati - certo, gli potevano essere forniti i dati delle pendenze in cassazione, ma non quelli presso le procure della Repubblica forse in vista di un ragionamento di incostituzionalità e, quindi, di violazione dell'articolo 3, proprio per porre i due uffici giudiziari nelle medesime condizioni di difficoltà. Questo elemento non è possibile rilevare; questo elemento non è stato offerto. Soltanto di fronte a una similitudine di difficoltà di due uffici giudiziari si può parlare eventualmente di una incostituzionalità della norma, perché il legislatore avrebbe affrontato e risolto il problema di un ufficio giudiziario e avrebbe lasciato invece l'altro ufficio nelle medesime condizioni senza il provvedimento "di aiuto" a smaltire il carico a smaltire il carico giudiziario. Questo è il problema. Allora abbiamo, per un verso, un provvedimento che va nella direzione di affermare il principio della durata ragionevole del processo. ricordo che vi è stato detto da un operatore del diritto che opera in quegli uffici giudiziari che, nella situazione attuale, servirebbero trent'anni per azzerare l'arretrato.

che vivono la medesima condizione di eccessivo carico giudiziario. Da qui scaturisce la straordinarietà dell'intervento.

come diceva il senatore Caliendo - che l'avvocato viene spogliato delle sue prerogative perché non partecipa alla camera di consiglio. Innanzitutto, l'avvocato scrive, in genere si parla di cause civili, e il principio generale che accompagna il processo civile è quello degli scritti, che vengono offerti all'organo giudicante. Non solo: è prevista anche la deroga, e cioè quando il presidente della sezione ritiene che quella vicenda meriti di essere illustrata dalle parti, queste hanno accesso alla camera di consiglio. Quindi, anche per detto verso, questo profilo mi pare essere del tutto inconferente. Rimane il dato:

tentar di affermare un principio costituzionale, noi perché non dobbiamo immaginare che venga data una proroga di un anno a coloro a coloro che stanno lavorando? Io credo che si offenda anche l'intera magistratura, perché un conto è fare un provvedimento *ad personam* al senatore Falanga, o al senatore Cuomo che è di fronte a me, e un conto è pensare di fare un provvedimento *ad personam* alla prima autorità giudiziaria, il primo presidente della Corte di cassazione. Non mi pare che queste siano

della violazione perenne e continua della ragionevole durata del processo. Chiunque adotti provvedimenti perché il nostro Paese possa garantire una durata ragionevole del processo, io lo sostengo. Il Gruppo AL-A sostiene questo provvedimento, ma sempre nell'ottica di condividere quei provvedimenti che apprezziamo. E questo è un provvedimento urgente e straordinario che noi non possiamo ostacolare. Noi non possiamo ostacolare un Governo che che adotta un provvedimento che vede affermare un principio di rango costituzionale. Non lo possiamo fare, a prescindere se facciamo o non facciamo, sosteniamo o no. Per le ragioni di diritto e di rango costituzionale, mi piacerebbe avere un confronto un po' più ampio con i senatori Caliendo e Gasparri proprio sul tema della incostituzionalità del provvedimento

senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2550,

La seduta è ripresa. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge sull'efficienza degli uffici giudiziari, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Per la discussione generale sulla fiducia, che avrà inizio alle ore 14,30, è stata ripartita un'ora e venti minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Le dichiarazioni finali di voto avranno luogo a partire dalle ore 15,50. Seguirà quindi la chiama alle ore 17,30. Subito dopo il voto di fiducia la seduta sarà tolta.

saranno eventualmente autorizzate a convocarsi al termine della seduta

alle ore 16, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senatrice Stefania Giannini, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: misure di sostegno pubblico alla ricerca e al sistema universitario; problematiche connesse all'avvio dell'anno scolastico, con particolare riferimento al reclutamento dei docenti.

*(CoR)*. Signora Presidente, credo che venga già spontaneo il commento. Basta guardare quest'Aula per esprimere che sentimento e che attenzione ci sono verso un provvedimento così importante. Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, che cosa si può dire di questo provvedimento se non denunciare ancora una volta il metodo che ormai caratterizza questa maggioranza, che ha in spregio regole e Regolamenti parlamentari, e constatare che spesso il metodo e il merito dei provvedimenti coincidono nel disprezzo del Parlamento e nel disprezzo per il Paese? Un disdoro che è il marchio di fabbrica dell'azione di questo Governo. Abbiamo tanto e troppo a lungo parlato in quest'Aula dei presupposti di necessità ed urgenza, della necessaria omogeneità delle materie che si vanno a regolamentare con decreto-legge, della mancanza ontologica di tali requisiti nei casi di riforme ordinamentali, dell'usurpazione da parte del Governo del potere legislativo all'organo costituzionalmente preposto ad esercitarlo e cioè al Parlamento. Ormai, poco convintamente, recitiamo e proponiamo pregiudiziali. Il mio Gruppo questa volta si è astenuto, ma apprezzo comunque la perseveranza dei colleghi che a questa funzione riescono ancora a dedicare il loro tempo. Una sorta di mantra, come un'insopportabile nenia che nessuno ascolterà. Ma, parafrasando la famosa frase sul giudice a Berlino: vivaddio, ci sarà un Colle in questa parossistica Capitale che vorrà prestare orecchio? O saremo costretti a scrivere la nuova fiaba del bell'addormentato sul Colle? Ma come si fa, nel perseverante vilipendio delle istituzioni, a chiedere di abbassare i toni? Ditemi, come si fa? A meno di non volere leggere nel richiamo del Presidente della Repubblica il famoso silenzio di Wittgenstein, e cioè quel silenzio... PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, come lei sa, il Presidente della Repubblica non è oggetto di discussione nell'Aula del Senato, quindi la prego di stare entro i termini *(CoR)*. Signora Presidente, io sto nei termini dovuti e i richiami sono pertinenti.

signora Presidente. A meno che il nostro Presidente della Repubblica in questo richiamo che fa non voglia rappresentare il silenzio di Wittgenstein, cioè quel silenzio che non è assenza di parola, ma è il limite estremo di essa. Ma, invero, mi sembra un richiamo troppo elitario per il livello culturale di questo Governo. Su questi incomprensibili silenzi intanto imperversa il Presidente del Consiglio, che ci ha soppressi, ha soppresso il dibattito parlamentare e, infine, ha rottamato una sola cosa: il cuore della nostra democrazia. Questo è l'ennesimo provvedimento che non solo presenta gravissimi *vulnus* costituzionali, peraltro rilevati anche dalla Commissione affari costituzionali, ma viene realizzato nel totale spregio dei problemi che creerà agli operatori del diritto, nella sua assoluta inutilità al fine di dare un valido contributo alla riduzione dei tempi della giustizia civile. E mi dispiace non sia presente in Aula il senatore Falanga, che stamattina ha tentato - anche lui - attraverso i suoi buoni uffici, di fare la foglia di fico su questo provvedimento. non dà risposte neanche alla richiesta di giustizia dei cittadini e, non ultimo, alla competitività e all'immagine del Paese a livello internazionale, a meno che le cene oltreoceano non servano anche a elevare lo *standing* del nostro sistema giudiziario. Dicevo non ultimo, perché, infine, il provvedimento in esame una mefitica funzione ce l'ha: paga il debito contratto con quei giudici imparziali che hanno permesso di licenziare il quesito referendario così come piaceva a questo Governo. Allora che dire? Non voglio urtare la sensibilità dei 160-180 senatori che costituiscono questa maggioranza (e dico 160-180 perché questa è una maggioranza variabile a seconda della questua del momento): non dirò che di marchette trattasi; dirò che con questo provvedimento si ricompensano quei giudici che hanno permesso di fare quel bottino. E non parlerò più, come sono stato invitato a fare, di postriboli; dirò che il Parlamento è ormai ridotto a mercato, dove, nella totale indifferenza di Presidenza e Quirinale, il mercimonio delle leggi è diventato consuetudine. leggi *ad personam* erano esercitazioni da principiante. Qui tocchiamo con mano il più sfacciato e ostentato disprezzo delle regole democratiche. Si è consumato un patto scellerato tra due poteri dello Stato in danno di un altro. Attenzione - mi rivolgo soprattutto alla Presidenza - che la spocchia e la superficialità con cui si accompagna questa pericolosa deriva portano necessariamente a non ragionare più con gli avversari politici, perché se si è contro le regole democratiche, se si calpestano e si occupano gli spazi dell'opposizione e se si è contro i dettami della Costituzione, alla fine, l'avversario politico diventa il nemico. Questo ha prodotto l'ottuso e pervicace disprezzo, da parte del Presidente del Consiglio, delle regole del gioco. Ha prodotto un Paese spaccato e diviso, dove i sentimenti di impotenza e di insoddisfazione covano astio e rancore, credo è naturale che sia. Allora non si può intervenire per dire di abbassare i toni. A noi non serve un sensale (e faccio notare, tra l'altro, che la parola «sensale» deriva dall'arabo e chi prende questa posizione di solito ha una parte in gioco). A noi serve un Capo dello Stato che riprenda e sanzioni chi si muove fuori dalle regole del gioco, un garante, insomma, come giustamente sostiene il Presidente di turno e come la Costituzione vigente non consiglia, ma impone. In questa Babele di regole, funzioni e procedure si inserisce questo scellerato provvedimento, che suggella e paga misfatti consumati in combutta tra Esecutivo e potere giudiziario. Pare ovvio che il Gruppo Conservatori e Riformisti, ancorato ai dettami costituzionali, voterà contro.

Come qualcuno ha detto, l'attuale maggioranza probabilmente è nata sulla scorta della convinzione che vincere le elezioni significhi essere proprietari delle istituzioni.

un decreto-legge che è viziato fin dal suo nascere dalla palese previsione di una discriminazione e da una palese violazione dei principi costituzionali dell'uguaglianza

Pensiamo dunque di dover cogliere l'occasione per dire che sicuramente quello al nostro esame non è un decreto che risolve i problemi della giustizia, non è un decreto che velocizza la giustizia, non è un decreto che semplifica la giustizia e, di certo, non si va verso quella che doveva essere la "grande riforma della giustizia". Ora possiamo fare una riflessione,

Quella riforma, signori, è stata preda di un ingorgo politico ed è caduta nella palude della politica, delle contraddizioni e delle divisioni politiche che avete al vostro interno.

Finché non arriveranno provvedimenti che inseriscano queste norme sulla giustizia, non voteremo mai a favore.

Signora Presidente, qui si continua con i decreti-legge, molti dei quali arrivano dalla Commissione giustizia. La collega Stefani ha appena parlato del senso di giustizia degli italiani, del carcere, dei reati.

ai contenuti del decreto-legge e con gli emendamenti siamo sicuri che la maggioranza di quest'Aula (maggioranza e opposizione) saprà modificarlo, a meno che non venga posta la fiducia. Ed ecco: è stata messa la fiducia.

per chiudere la discussione perché era vitale che il martedì questo decreto-legge fosse convertito. Siamo a mercoledì. Certe volte sembra veramente di essere dentro una commedia all'italiana, ad una dissociazione

che il decreto-legge si applichi anche ai magistrati della Corte dei conti, a quelli del Consiglio di Stato, a quelli contabili e amministrativi. Quanti sono i magistrati della Corte dei conti e del Consiglio di Stato a cui si applica questo decreto-legge? È una foglia di fico forse? Qualcuno si vergognava del fatto che fosse applicabile soltanto ad alcuni magistrati della Cassazione? Il collega Di Maggio ha parlato di un premio, di un *do ut des*. Sicuramente c'è anche da domandarsi: perché il premio è graduato? Lo sapete che c'è chi, come il primo presidente, viene prorogato di un anno (doveva andare in pensione il 1° gennaio e viene prorogato al 31 dicembre), e altri, invece, di quella piccola lista, hanno una proroga di soli tre mesi? Non soltanto, quindi

hanno posizioni apicali sul territorio e avrebbero avuto lo stesso diritto, ma, anche all'interno dei beneficiati, dei premiati, c'è stata una graduatoria: sono beneficiati di più alcuni, che staranno un anno in più rispetto al previsto, rispetto ad altri,

Secondo quello che ha detto la prima sezione civile, precostituita ad arte, lo può fare e lo stava per decidere anche la sesta sezione. Ma perché, in uno Stato di diritto, visto che l'ordinamento prevede questo per l'unicità della giurisdizione, il primo presidente il primo presidente della Cassazione, visto che il procuratore generale glielo ha chiesto per iscritto in udienza, decine di senatori e deputati lo hanno scritto e il Parlamento ha stralciato la *stepchild adoption*, non demanda la decisione Perché non fa decidere le sezioni unite che per legge devono farlo? Perché ci manda una lettera, ironica o di presa in giro, in cui dice che «per prassi» fa decidere la sezione interessata? Per prassi fa decidere la sezione interessata, quando la responsabilità è per legge del primo presidente?

volete che venga confermato il bicameralismo, sia pure con funzioni diverse tra Camera e Senato delle Regioni? Italiani, volete che ci sia un risparmio sulla politica dello 0,0005 per cento, così come definito dalla Ragioneria dello Stato?». È passato un altro testo alla Cassazione. E allora, il collega Quagliariello si è posto il problema: c'è forse una qualche relazione tra questo premio che viene dato e quel tipo di comportamento? Non è che la politica del Governo incida sui magistrati? Altro che polemiche sul «ci si difende nei processi, non dai processi». Ricordo che nel 1994-1996, due famosi esponenti di Forza Italia, di cui non faccio il nome, discutevano tra di loro, uno bravo, diligente, preparava tutte le comparse e l'altro che gli diceva: «Ma perché ti dai tanto da fare?

per dare questo premio. Alcuni colleghi si sono chiesti se siamo in uno Stato di diritto o se siamo ormai in un rapporto in cui il Governo fa strame del Parlamento, in cui gioca con la magistratura, per ottenere decisioni Non sto parlando qui del merito delle questioni. Non sto dicendo se l'adozione di un bambino da parte di una coppia *gay* o l'odiosa pratica dell'utero in affitto siano

Ma vi rendete conto di quello che sta capitando? Non voglio parlare del merito, ma del metodo. Qui si continua a violare la legge e si continuano a premiare quelli che violano la legge. E se è il primo presidente della Cassazione a violarla, è ancora peggio! È per questo che abbiamo scritto anche al Capo dello Stato: qualcuno deve intervenire

si presenta al Parlamento per chiedere la fiducia. Cosa avviene sotto il profilo squisitamente costituzionale? Avviene un controllo da parte del Parlamento sul Governo. Altra ipotesi: il Governo in carica ha una legge e ritiene di porre la fiducia su quella legge. Si inverte la questione, perché è il Governo che che viene a chiedere al Parlamento e controlla (adesso il Governo e non più il Parlamento) la sua maggioranza. Sono due questioni, due momenti,

non abbiamo dato la fiducia al presidente Renzi quando, composta la squadra, è venuto qui in Parlamento a chiedere la fiducia, sulla base di un

con un proprio programma e noi (parlo dei miei colleghi di Gruppo che in quel momento erano in altre forze politiche, in particolare in Forza Italia) al Parlamento, non lo condividemmo e quindi non votammo la fiducia. Nel corso dell'espletamento del mandato di Governo mandato di Governo sono state discusse alcune leggi che non erano in quel programma, ma che erano da noi condivise.

e quindi era giusto che la votassimo. L'abolizione dell'IMU è stato un cavallo di battaglia del presidente Berlusconi e abbiamo votato quel provvedimento. Ciò significa che la fiducia che oggi ci apprestiamo a dare è limitata esclusivamente a questo provvedimento.

perché vi sia un'ipotesi di incostituzionalità, occorre che vi sia una legge che su due situazioni identiche identiche disponga diversamente per l'una e per l'altra. Colleghi, abbiamo 105.000 procedimenti civili pendenti in Cassazione.

Se vi sono provvedimenti che vanno nella direzione di ridurre questo carico giudiziario per l'affermazione di un principio costituzionale, mi domando come si possa sanzionare il provvedimento con l'incostituzionalità.

ne abbiamo prova - il medesimo carico giudiziario e si interviene lì dove c'è quella situazione, per porre rimedio a una violazione di norma costituzionale. Tutto qui. Noi voteremo la fiducia e cosa significa? Lo abbiamo detto in varie occasioni e in vari modi: votare la fiducia sul provvedimento, vuol dire

noi votiamo la fiducia sui provvedimenti che riteniamo di poter condividere. Domani, se il Governo ponesse la fiducia su un provvedimento che noi, da liberali, potremmo verificare che di liberale non ha nulla, non voteremo la fiducia. Questo è il modo più corretto di adempiere al mandato parlamentare.

che dispone la proroga dei vertici della Cassazione e che va a rivisitare il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione e lei parla di *stepchild adoption*. Mi domando: che c'entra? Dire no, sempre e a prescindere! E sentiamo l'illustre collega Stefani, della Lega Nord, parlare dei furti negli appartamenti. Ma scusate, che cosa c'entrano queste cose qui? Parliamo del provvedimento che stiamo esaminando. Non volete approvarlo? Bene. Volete che permanga questo carico giudiziario in Cassazione di oltre 105.000 non riuscirà, con questo provvedimento, a smaltire quel carico? Può darsi, però io apprezzo il tentativo, apprezzo la volontà, comunque, di intervenire. E non si parli di provvedimenti *ad personam*. Non si conviene, quando si parla, non già di Ciro Falanga o del Milo, ma del primo presidente della Corte di cassazione, la massima autorità della giustizia del nostro Paese, che non ha di certo bisogno di rimanere ancora un anno in servizio. Anzi, forse gli stiamo chiedendo un piacere, che lui probabilmente ci farà. Si sta ponendo a disposizione del suo Paese per risolvere o tentare di risolvere i problemi della giustizia. Io non sono, senatore Calderoli, un anatomopatologo

Governo, invitandovi ancora una volta, ove mai - e lo comprendo - non vi piaccia, ad accettare, perché dovete accettarla, la nostra lezione di democrazia.

mi dispiace che gli studenti e gli insegnanti siano andati via, perché una lezione di democrazia che il Senato impartisce a noi, per loro poteva essere particolarmente interessante. sono sempre attento alle lezioni, caro senatore Falanga, e ho capito che ella ha detto che questo decreto-legge è un buon decreto-legge e quindi AL-A, il Gruppo costruito da Verdini per soccorrere il Governo Renzi, non ancora accolto in maggioranza, in questo caso lo voterà. Ma chiedo a tutti noi: perché, se questo decreto-legge è così forte, condivisibile e senza problemi, è stata posta la fiducia? Perché non farlo approvare rapidamente dall'Assemblea? Devo dire che ho apprezzato lo *charme* con cui la Ministra per i rapporti con il Parlamento ha chiesto l'ennesima fiducia. Ma, se fosse ancora in Aula (cosa che non è), vorrei chiederle un piccolo chiarimento, cioè vorrei chiederle cosa sia cambiato negli ultimi venti giorni. Infatti, signora Presidente, come lei ricorderà, il 28 settembre il presidente del Consiglio Matteo Renzi, a proposito di un altro provvedimento, più generale, ha detto tendenzialmente si sentiva di escludere la fiducia sulla riforma della giustizia in discussione al Senato, perché si sarebbe trattato, in sostanza, di un atto ostile nei confronti dell'Associazione nazionale magistrati. Anche questo provvedimento riguarda quella funzione (la magistratura, l'esercizio del processo), che è una funzione per la quale la Costituzione ha previsto una forte autonomia

che le discuta in modo trasparente, che si dia un senso a quell'idea che il Parlamento legifera in nome del popolo e rappresenta il popolo. Allora, diciamo chiaramente che la ragione per cui la ministra Boschi ha chiesto la fiducia è che alcuni emendamenti critici,

che è tutto legittimo, perché il Governo ha la maggioranza. È vero, il Governo ha la maggioranza, però dobbiamo chiederci, dopo tre anni, che maggioranza abbia questo Governo. In parte, è una maggioranza che deriva dal premio spropositato previsto da una legge elettorale veniva chiamata volgarmente Porcellum e che è stata dichiarata incostituzionale. In parte, viene dall'acquisizione dei consensi di parti del principale partito partito di opposizione, che sono state sedotte dalla politica trasformista del Governo Renzi. Una maggioranza siffatta impone la sua legge per fiducie, sistematicamente esautora le Commissioni e quindi umilia l'Aula, perché in Aula non si discute: in Aula si vota. Vedete, l'assenza dei senatori qua dentro non è dovuta a un impertinente demone meridiano che li ha presi

ne abbiamo viste tante. Ricordo alcune di queste gravissime violazioni del diritto parlamentare. Non parlo del Presidente della Repubblica, signora Presidente, al quale bisogna riferirsi il meno possibile da queste Aule. Parlo però del diritto parlamentare. Ne ricordo una, che mi è ancora della discussione della legge di riforma sulla scuola, la Commissione istruzione di questo Senato era orientata a cambiare profondamente il provvedimento. Ad un certo punto, persino il Presidente del Consiglio si era convinto che fosse utile cambiare quella riforma e lo disse in una trasmissione pubblica da Vespa. però ci ha ripensato; alcuni senatori e alcuni deputati sono andati da lui dicendogli che ci avevano messo la faccia, il Presidente del Consiglio ha visto l'occasione per passare in forza, ha tolto il provvedimento alla Commissione, che non ha potuto discuterlo, e l'ha fatto passare con la fiducia. Questo è il riformismo del Governo Renzi. Ma io mi chiedo: è un buon riformismo? Certo, rompe le uova del diritto parlamentare, delle tradizioni e, secondo me,

le ha dato un cinque scarso, mentre, guarda un po', ha difeso tutti quegli insegnanti umiliati, deportati, messi sotto un controllo amministrativo

non aveva accettato di andare fuori perché aveva famiglia e magari perché era bravo e pensava di essere chiamato a casa sua, è rimasto completamente per strada. Gli insegnanti vengono salvati da quel sondaggio di opinione. Ma vorrei dire un'altra cosa. Abbiamo visto tutti quale successo abbia avuto il nostro Presidente del Consiglio a Washington; attualmente, come italiano, sono contento di quelle pacche, di quegli abbracci,

oggi un grande vignettista su un giornale che non è proprio un foglio dell'estrema sinistra, il «Corriere della Sera», immagina che Renzi sia caduto dalla sedia durante quella cena di Stato perché gli erano arrivate le notizie dall'Italia. Le notizie dall'Italia dicono che le assunzioni stabili

*jobs act* è che sono aumentati fortemente i licenziamenti per giusta causa, ora che non c'è più l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Il *jobs act* è stato un fallimento molto più grave della buona scuola, perché non ha avviato neanche quelle politiche attive del lavoro lavoro che ci sono in Germania, per cui il lavoratore disoccupato viene vessato fino quando non accetta un lavoro, che sono l'altra parte di una politica di questo genere e che sono auspicate dalle stesse istituzioni che plaudono *obtorto* *collo* alle riforme di Renzi. Neanche questo vi è stato nel *jobs act*; vi è stato solo un rimettere i nostri ragazzi all'anarchia del mercato, perché il riformismo del nostro Governo è casuale, confuso e strumentale. È casuale, perché le ragioni delle riforme sono legate all'andamento dell'opinione pubblica: a un certo punto si capisce che un tema è popolare e, allora, via. Avete visto il provvedimento sull'abolizione di Equitalia naturalmente, per lisciare dalla parte del pelo un pezzo del popolo italiano. Questo è populismo, ma non si può parlare di populismo perché molti colleghi pensano sia un insulto destinato alle opposizioni; invece vi è un fortissimo populismo di Governo, anzi spesso il populismo il populismo è soprattutto di Governo. È confuso, perché le riforme contengono cose che non riescono a stare insieme. Pensate alla riforma costituzionale,

ad affermare la propria presa sulla maggioranza e sulle istituzioni e il proprio mantenimento al Governo. Questo è ciò cui stiamo assistendo: è un quadro davvero desolante. Da questo punto di vista, penso che, con con costanza, dobbiamo far battaglia e chiedere conto al Governo tutte le volte, anche se siamo stanchi, anche se ci sembra inutile. Presidente del Consiglio, perché lei aveva detto che non si sarebbe mai sognato di mettere la fiducia su una questione che riguardava la giustizia e oggi ci troviamo a votare la fiducia

a nome del Gruppo Area Popolare (Nuovo Centrodestra-Unione di Centro), esprimo parere favorevole sull'Atto Senato 2550, di conversione in legge del

sappiamo già essere incostituzionale, non meno di quella che ha portato gli attuali parlamentari della Camera e del Senato a sedere qui; da una maggioranza parlamentare che ormai ha già da tempo cestinato l'articolo 77 della Costituzione in tema di decretazione d'urgenza; da una maggioranza parlamentare che forza i lavori nelle Commissioni parlamentari, nell'applicazione del Regolamento d'Aula, nelle sostituzioni dei propri membri nel corso dell'*iter* della riforma costituzionale, che continua ad apporre un numero di questioni di fiducia di cui abbiamo perso il conto (ormai non so quante siano); da una maggioranza così, che si muove con una protervia e un'aggressività che cercano di essere nascoste dal decisionismo renziano, evidentemente non siamo sorpresi dall'esito di oggi, che pure avevamo paventato questa mattina, ossia che questa legge di conversione di un decreto-legge termina con l'apposizione della fiducia.

Forse potremmo essere più utili fuori da questo palazzo, magari facendo informazione o controinformazione. Però ogni volta troviamo i motivi per riuscire a svolgere il nostro ruolo di opposizione con le armi a nostra disposizione e per lasciare comunque negli atti del Senato testimonianza di quello che diciamo e delle cose che facciamo. Anche perché

non tanto il sottoscritto ma colleghi ben più autorevoli di me, hanno lasciato traccia negli atti. Della questione degli articoli 5 e 10 del testo già si è discusso ampiamente questa mattina in sede di illustrazione delle pregiudiziali di costituzionalità. Qui c'è un grande fraintendimento che anche nelle risposte del relatore e di altri esponenti della maggioranza si è fatto finta di ignorare. Il problema della discriminazione creata dalla misura

infatti c'erano emendamenti in quella direzione - semplicemente prorogando tutte le figure magistratuali (civili, amministrative, contabili e tributarie)

lascia aperta l'ipotesi del sospetto, che qui è stato avanzato da diversi colleghi che sia una norma mirata, che possa addirittura essere una sorta di merce di scambio, anche in relazione a recenti determinazioni della Suprema corte in tema di legittimità dei quesiti di un certo *referendum* costituzionale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. A noi non piace vivere nel sospetto. Ecco perché Ecco perché i profili di illegittimità costituzionale in relazione ai suddetti due articoli potevano superarsi con una norma che tenesse conto di quanto il relatore e la maggioranza ci avevano rappresentato: c'è un carico gravoso in Corte di cassazione;

Devo anche dire che ho ascoltato attentamente - peccato che adesso sia impegnato in una conversazione telefonica - il Presidente della Commissione giustizia, che è persona da tutti estremamente stimata per le proprie competenze anche di natura giuridica.

evidentemente non ha fatto una lettura abbastanza approfondita del testo, perché l'ho sentito sostenere tesi tranquillizzanti che sono smentite dalla norma. La cosa che noi denunciamo con riferimento alla modifica degli articoli del codice di procedura civile relativa al procedimento dell'inammissibilità dei ricorsi non attiene al fatto che sia una camera di consiglio.

nel testo che state per approvare con la fiducia non vi è più la possibilità di essere ascoltati in camera di consiglio; attenzione, non c'è più. Oggi c'è nel codice di procedura civile (articolo 380-*bis* e seguenti). Qui non c'è più. un'altra cosa che viene meno, su cui pure non vi è stata alcuna replica. Nel caso di dichiarazione di inammissibilità, oggi le parti sono rappresentate dagli avvocati, ma ricordiamoci che dietro gli avvocati ci sono dei cittadini. C'è qualcuno che in questo Paese ancora crede che la giustizia possa essere amministrata in maniera terza e imparziale. Oggi il relatore della Corte di cassazione deposita in cancelleria una relazione con la concisa concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare una pronuncia di inammissibilità e successivamente viene fissata l'udienza camerale alla quale oggi le parti, se lo richiedono, possono partecipare, mentre domani non più. della concisa esposizione delle ragioni che prefigurano una possibile inammissibilità scompare nel nuovo testo dell'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile come previsto nel disegno di legge.

di un ricorso o atto difensivo. L'approvazione di una tale norma è la morte di ogni processo giusto ed equivale alla negazione di poter far valere davanti a un giudice imparziale i propri interessi legittimi e diritti soggettivi. Questa previsione, che obbliga le parti a contingentare le proprie difese in una misura predeterminata di pagine, è ridicola, incongrua e gravemente contraria alla Costituzione. È ridicola perché non si può ridurre l'attività defensionale forense a una mera computazione di caratteri, margini e interlinee. È incongrua perché non tiene conto che vi sono liti che richiedono un'ampia trattazione e altre meno e che, nel primo caso, tutta la difesa possibile deve essere spiegata ed esercitata. Soprattutto, è gravemente anticostituzionale,

altresì, in modo non meno scandaloso, l'articolo 24 della Costituzione, risolvendosi la misura in un'effettiva e incomprensibile violazione del principio di tutela dei diritti e degli interessi legittimi.

noi diciamo no. Ancora una volta, anche se non fosse stata apposta la questione di fiducia, avremmo votato no, per i motivi che abbiamo cercato di illustrare.

Salutiamo e diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Medi-Livatino» di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti. ha facoltà. PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, credo che questa mattina, nell'illustrazione della pregiudiziale di costituzionalità, il senatore Caliendo abbia espresso, in termini estremamente chiari, la posizione del Gruppo Forza Italia. Non vi era una contrarietà di principio al provvedimento in esame, ma vi era una contrarietà al provvedimento così come esso era stata formulato. Vi era il tentativo da parte di Forza Italia - e, devo dire la verità, anche da parte di altri Gruppi di opposizione - di modificare il decreto-legge senza snaturarlo, ma al solo fine di evitare la possibile aggressione futura in sede di Corte costituzionale. Avete burocraticamente bocciato la pregiudiziale di costituzionalità, ma - devo dire la verità - non so per quali motivazioni, perché quelle che sono state fornite non mi sembrano né adeguate, né consone. Non è stata spesa una sola parola circa il fatto che l'articolo 1-*bis* sia stato inserito alla Camera dei deputati in totale disomogeneità di materia, nonostante la Corte costituzionale, con riferimento alla cosiddetta legge Fini-Giovanardi, fosse già intervenuta bocciando talune norme per incostituzionalità, proprio perché inserite in termini disomogenei rispetto al decreto-legge. Non avete speso alcuna parola sull'articolo 7, comma 7, ovvero sulla sproporzione di rappresentanza che create all'interno del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Infine, vi siete soffermati, leggendo solo quello che vi faceva piacere leggere, sull'annoso problema dell'articolo 5, ovvero sulla proroga dei magistrati.

Mi permetto di dire che il problema che ponevamo e che risulta in termini chiari dai dati è completamente diverso. Il problema non è che sono pendenti 106.000 cause davanti alla Corte di cassazione in sede civile, ma che in questo anno, in cui si è già registrata la prima proroga, vi è stato un aumento di queste cause; il che dimostra in maniera inequivocabile che la proroga come misura tampone non non ha nessuna capacità di ordine strutturale ed è destinata a fallire rispetto all'obiettivo prefissato, che è l'abbattimento delle pendenze. Il senatore Falanga dice che siamo destinati, per anni e anni, a non osservare il principio della ragionevole durata del processo in ragione delle pendenze che ci sono in Cassazione. Ciò vuol dire, sottosegretario Migliore, me lo spieghi bene - che per anni e anni, ogni anno, farete una proroga, perché per anni e anni ci sarà la situazione della pendenza? Non sarebbe forse più logico mettere da parte le misure tampone e intervenire finalmente con misure strutturali? L'amara realtà di ciò che stiamo discutendo oggi è però l'ennesimo fallimento della politica del Governo, in questo caso nel settore della giustizia. Quando nel 2014, forse giustamente, a settant'anni l'età di pensionamento dei magistrati, vi abbiamo detto in tutte le salse che questa vostra iniziativa, se non fosse stata accompagnata da misure transitorie, che garantissero una certa gradualità, avrebbe comportato notevoli difficoltà nell'efficienza dei uffici giudiziari. Ci avete detto di no: *hashtag «*lavoltabuona». Di lì a un anno avete fatto la prima proroga, proroga, ma era una proroga generale perché riguardava tutti gli uffici direttivi e semidirettivi della magistratura; aveva un senso, ma di lì a un altro anno avete disposto una successiva proroga e la situazione non è cambiata, anzi è peggiorata, e invece di ripetere la proroga del 2015 così come era stato segnalato in taluni emendamenti, credo sia del Movimento 5 Stelle che di Forza Italia, vi siete ostinati a una proroga assolutamente parziale che riguarda solo 13 persone della Corte di cassazione. La necessità di una proroga c'era, ma di una proroga che avesse come destinatari non solo 13 persone, ma l'intero comparto degli uffici direttivi della magistratura. Oppure volete venirci a dire che, grazie a queste 13 persone, di qui a un anno la pendenza sarà completamente abbattuta?

Io sono rimasto dispiaciuto e per certi versi anche amareggiato per parte del dibattito che si è sviluppato questa mattina.

con particolare riferimento alla parzialità dell'intervento, invece che alla generalità che tutti quanti (noi di Forza Italia per primi) auspicavamo. Hanno sostanzialmente pronunciato parole di forte critica nei confronti degli alti vertici della magistratura, parole che non sarebbero state mai pronunciate se il provvedimento fosse stato identico a quello di un anno fa o se avesse avuto un contenuto più generale e non si fosse nascosto, sottosegretario Migliore, dietro il ridicolo paravento di una pendenza. Avete consentito che il prestigio della magistratura

venisse additato all'opinione pubblica come il mandante occulto di questo provvedimento.

Non si varano delle norme ordinamentali ancorandole a una fasulla motivazione, perché poi la conseguenza è esattamente quella che oggi abbiamo visto in quest'Aula e di cui domani troveremo traccia sui giornali. Questo è nella realtà il delitto più importante che voi avete commesso e non sotto il profilo tecnico (ormai da tanti anni sono abituato al cinismo con cui le questioni tecniche vengono trattate in quest'Aula); il vostro è un errore enorme sotto il profilo politico. Questo decreto-legge, che già sui giornali viene indicato come legge Canzio, come legge Canzio, va a toccare l'immagine di un grandissimo magistrato, uno dei migliori magistrati che l'Italia ha avuto. Vedete, potrei continuare, ma nella realtà non ne ho più voglia perché non ha senso continuare. Il senatore Lumia, con un'approssimazione alla verità che lo contraddistingue, nel suo intervento di oggi ha detto che in Commissione vi è stato un approfondito dibattito: dieci ore.

questioni così importanti come quelle contenute all'interno del decreto-legge? Si può sceverare il permanere dei magistrati, l'alterazione del consiglio di presidenza? Non ci avete consentito di votare, con un *blitz* - devo dire la verità che non riesco neanche ad appellare. È per questo, signora Presidente, signori colleghi, che il Gruppo Forza Italia non parteciperà al voto. Vi siete

Ci sarete voi a dover mostrare la faccia quando la Corte costituzionale lo decapiterà. Per questo non parteciperemo al voto. Faccio l'ultima considerazione, Presidente. Ho letto l'intervento della senatrice Lo Moro. Senatrice, lei ha un grande coraggio. Io condivido tutto quello che ha detto, però mi permetta di dirle una cosa: noi non partecipiamo al voto, il che evidentemente, ove mai fosse necessario, rende scontato l'esito del voto

negoziandola con la vostra coscienza? Quella coscienza, senatrice Lo Moro, che lei ha dichiarato in termini molto chiari. Ne approfitto per dire che questo provvedimento può passare solo con la fiducia, perché il Governo sa che rischierebbe fortemente sugli articoli, 5, 7 e 10. Abbiate il coraggio, come lo avete avuto nel fare queste dichiarazioni, di non votare la fiducia.

è ormai risaputo che, quando si affrontano temi che hanno per oggetto la riforma della giustizia, il percorso del Parlamento diventa difficile: il confronto tra la maggioranza e l'opposizione normalmente deraglia, spesso si utilizzano argomenti - come tutti i colleghi hanno potuto sentire in quest'Aula - che non attengono al merito, in questo caso, del decreto-legge. Si è parlato molto di riforma costituzionale; si è parlato molto addirittura di legge elettorale, si è discusso di argomenti che non hanno alcuna attinenza con la portata normativa descritta e presentata in tutti gli articoli. A nostro avviso, signora Presidente, onorevoli colleghi, la riforma della giustizia comunque deve andare avanti. È un percorso difficile, pieno di trappole, accidentato, caratterizzato da profonde divisioni, aperto anche a tutte le strumentalizzazioni, spesso anche a quelle che si presentano nelle forme più teatrali possibili, come abbiamo potuto ascoltare adesso. problema di complessità e delicatezza. Ebbene, nonostante queste caratteristiche, la responsabilità di andare avanti ce la assumiamo tutta. Non abbiamo paura, finalmente, in questa legislatura, di procedere verso la riforma della giustizia, di farlo con diversi provvedimenti, facendo in modo che tutto il Parlamento partecipi al confronto.

Quella teatralità cui facevo riferimento a un certo punto si tradisce. Dire infatti che si sono dedicate dieci ore di discussione a questo provvedimento, un decreto-legge che volutamente è stato rinviato a lunedì di questa settimana (perché ci è stata richiesta ben una settimana di tempo per presentare degli emendamenti), tradisce appunto lo stile, il rigore e la serietà delle osservazioni critiche che sono state fatte. Nessuno scandalo. In questo provvedimento, cari colleghi, sono contenuti diversi punti che partono da un dato oggettivo che non si può nascondere e che non è stato

Cari colleghi, non vi troverete di fronte un decreto-legge che fa la scelta, in quel caso sì riduttiva, banale e puerile, di prorogare per un anno anno i vertici apicali della Cassazione per chiudere definitivamente quel contenzioso. Avete di fronte un insieme di norme che sono, anche nella loro

Per la prima volta, dopo tanti anni di discussione, si fa la scelta di utilizzare quel patrimonio e quell'elevato numero di magistrati di merito addetti al massimario per dare una mano ad abbattere questo contenzioso; si fa in modo improvvisato, ma rispettando le tabelle di organizzazione della Corte e le esigenze dell'ufficio del massimario. cari colleghi, si fa in modo, con un intervento omogeneo con le caratteristiche del decreto, di sveltire quella che viene chiamata la trattazione in camera di consiglio dei procedimenti civili, che si svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte; e si propongono anche delle modifiche alla procedura del cosiddetto filtro in Cassazione.

norme sulle droghe pesanti e sul recupero dei tossicodipendenti. Ricordo che il decreto-legge con il quale si compì quella incursione corsara riguardava misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali. Qui invece, cari colleghi, stiamo parlando di misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. Più omogeneità di questa è difficile trovarne.

di un particolare snodo della giustizia del nostro Paese, quelli di sorveglianza. Si interviene, cari colleghi, ancora per diversi articoli sulla giustizia amministrativa e, in particolare, sul processo telematico utilizzato nel processo amministrativo. Ecco perché

le ingiurie e gli insulti verso chi invece, come Governo e maggioranza, propone il via libera a questo decreto-legge. È troppo facile, troppo scorretto; bisogna imparare a rispettare le alte cariche delle istituzioni, a non inserirle nel gioco delle polemiche del Parlamento e della politica e, quando lo si fa, bisogna chiedere scusa e non scaricare agli altri questa responsabilità. Cari colleghi, ci aspettano altre tappe importanti della riforma della giustizia, in testa la riforma del processo civile, di quello penale penale e di tanti altri aspetti importanti che incidono sul buon andamento, sulla velocità e la capacità nel nostro Paese di fornire ai cittadini un servizio moderno e avanzato. È chiaro che la polemica ci accompagnerà e ci sarà sempre. Si è svelato facilmente, attraverso alcuni argomenti molto seri e ben strutturati, a partire da quelli del Presidente, il valore e la coerenza costituzionale del decreto-legge. È chiaro che, di fronte alla complessità, ci potevano essere altre soluzioni. Le abbiamo discusse ed erano tutte legittime e valide, ma, con un gioco strumentale cosa si prende una di queste valide soluzioni e si pensa di utilizzarle come clava contro le altre, che hanno la stessa legittimità e che hanno la stessa possibilità di incidere su quel provvedimento. Ecco perché mettiamo da parte le strumentalizzazioni e diciamo al Governo, alla maggioranza e all'opposizione di andare avanti. Il merito prevarrà; la stagione delle divisioni - quelle sì - cattive quelle sì - cattive e legate alle leggi *ad personam* sono alle nostre spalle. Procediamo e andiamo avanti perché la riforma della giustizia è un dovere che ci appartiene e poi a questo dovere ci appelliamo e non ci rinunciamo.

con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Invito ora il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Fasiolo.

Cucca,

Pinotti,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

alla ricerca e al sistema universitario; problematiche connesse all'avvio dell'anno scolastico, con particolare riferimento al reclutamento dei docenti. **Ripresa della